Comunico che, in data 3 settembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: «Onorevole Presidente, informo la Signoria Vostra che con decreti del Presidente della Repubblica in data odierna, adottati su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri,

Signor Presidente, ci avviamo alla votazione del disegno di legge di conversione dopo un'attenta discussione, che ha visto davvero un lavoro intenso, il confronto fra tutti i Gruppi parlamentari e il dialogo con il mondo produttivo, accademico, sindacale, delle professioni e dell'associazionismo. Abbiamo infatti acquisito, anche in relazione alla complessità e alla varietà dei temi trattati, circa 90 contributi scritti da parte di tutte le categorie di esperti, che abbiamo audito nelle Commissioni congiunte 1a ed 8a, portando avanti il lavoro con il contributo attivo e fattivo del Governo e il supporto costante degli Uffici del Senato e dei Gruppi parlamentari, cui rinnovo il ringraziamento. Nonostante si sia dovuto procedere un po' a tappe forzate, per la coincidenza dell'esame di altri provvedimenti, le scadenze connaturate al procedimento di conversione e l'ampia estensione dei temi trattati, credo possiamo affermare con soddisfazione di aver svolto un esame attento, che non solo ha contribuito a migliorare significativamente il testo, ma che ha fornito a tutti noi elementi di conoscenza e di riflessione per il prosieguo dell'attività legislativa. L'importanza e l'utilità del lavoro svolto sono state riconosciute, pur nell'inevitabile differenza di accenti e di opinioni, anche da molti degli interventi dei colleghi, sia di maggioranza che di opposizione. Come ho già avuto modo di dire in sede di relazione, era chiaro fin dall'inizio che il novero delle problematiche da affrontare era ampio e reso ancora più urgente della complessa situazione che stiamo vivendo. Era evidente - lo dico ad alcuni colleghi, che pure hanno richiamato diverse questioni meritevoli di attenzione - che un provvedimento come questo, che già contiene norme disparate ed eterogenee, non può né poteva rispondere ad ogni e qualsiasi problematica. D'altro canto - mi consentirete la riflessione - molte misure essenziali per la modernizzazione della pubblica amministrazione, per la semplificazione dei procedimenti, per la razionalizzazione e l'adeguamento della disciplina dei diversi settori, mai avrebbero potuto trovare attenzione ed accoglimento se non nell'ambito di un provvedimento dichiaratamente di natura ordinamentale, di un intervento che persegue esplicitamente e direttamente questi scopi. D'altronde, per citare uno degli aspetti del decreto-legge che ci accingiamo a convertire, aver riconosciuto la dimensione della cittadinanza digitale, delle opportunità per cittadini ed imprese di interloquire sempre ed efficacemente con la pubblica amministrazione mediante canali telematici è un'esigenza maturata nel tempo, che l'emergenza legata alla pandemia ha portato allo scoperto in tutta la sua urgenza. Non possiamo esimerci dal riconoscere un'esigenza del genere, a pena di determinare una sempre più profonda scollatura fra una società e un tessuto economico, per i quali gli strumenti digitali sono ormai parte integrante della vita quotidiana, e un'amministrazione pubblica, che nonostante gli sforzi e le innovazioni introdotte, non è ancora del tutto attrezzata a gestire i procedimenti nella loro interezza nella forma digitale,

Proprio su questo punto si gioca in gran parte la sfida della ripresa economica e della competitività del sistema Paese, che non potrà mai rialzarsi e reggere il ritmo del resto d'Europa senza garantire strade, porti, ferrovie, autostrade,

fino all'impiantistica sportiva, significa liberare energie produttive e impiegare un'immensa massa di risorse bloccate dall'inerzia della burocrazia, dal gioco dei veti, da un ricorso spesso improprio a contenziosi davanti alla giurisdizione amministrativa. una massa di risorse e di interventi che possono rappresentare già di per sé uno *shock*, specie per quei sistemi economici locali che già languivano prima della grande crisi e per i quali avviare i lavori significa, sia generare nell'immediato occupazione, che dotarsi di strumenti che ne consentano uno sviluppo duraturo. A quanti rilevano i limiti di un provvedimento ordinamentale è facile rispondere che a poco o nulla serve stanziare risorse per l'una o per l'altra ottima finalità, per una o per un'altra infrastruttura strategica o programma di investimento, se poi quelle risorse non si riescono effettivamente a spendere, se poi quelle ottime progettualità rimangono incagliate in procedure irrazionali, farraginose e insensate. A ben guardare, eliminare gli ostacoli e semplificare le procedure per le infrastrutture, come per l'iniziativa privata, restituisce alla politica e alle istituzioni un potere di scegliere e orientare che troppo spesso, nei fatti, stato distorto e imbrigliato, attribuendo impropriamente poteri di veto a troppi soggetti che non necessariamente rispondono all'oggettivo interesse pubblico. Si tratta anche di contribuire a ridisegnare il ruolo dell'amministrazione, restituendo un quadro di maggiore certezza di competenze e responsabilità, a partire dalla dirigenza, per arrivare ad ogni ufficio e servizio, dove il cittadino deve poter trovare interlocutori attenti che diano risposte in tempi certi, secondo procedure trasparenti e imparziali, perché è proprio la tendenza all'inerzia, favorita da un quadro poco chiaro delle norme, la patologia che già affliggeva il sistema Italia: un circolo vizioso che si autoalimenta e che deve essere spezzato.

Alleggerire perciò il percorso di realizzazione delle infrastrutture, semplificare i procedimenti amministrativi, modernizzare la disciplina di molti settori, dare garanzia a cittadini e imprese di un rapporto trasparente, veloce e digitale con la pubblica amministrazione sono le sfide cui siamo e saremo ancora chiamati, le sfide alle quali iniziamo a dare una risposta concreta e forte con questo provvedimento. È necessario e urgente pertanto procedere con decisione, anche con ulteriori provvedimenti, nel processo di semplificazione amministrativa, al fine di rendere più comprensibile e snello il funzionamento della pubblica amministrazione. Per questo, in conclusione, non prima di aver rinnovato a tutti il ringraziamento per il proficuo lavoro svolto, auspico che questo spirito e questa direzione di marcia possano ispirare l'ancora grande lavoro che abbiamo davanti, perché un Paese più semplice è un Paese più giusto, cui noi legislatori dobbiamo offrire gli strumenti perché possa rialzarsi e riprendere a correre, finalmente libero dai troppi lacci e vincoli che mortificano le migliori idee, intelligenze, capacità e progettualità dell'Italia.

Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato con attenzione gli interventi, in molti dei quali è stato sottolineato il quadro generale che da mesi ha stravolto i lavori parlamentari e la vita di milioni di italiani e che ha determinato la nascita di questo decreto-legge, nel quale sono inseriti elementi di non poco conto. Tornare alla normalità non è e non sarà facile, anche perché l'emergenza sanitaria non può essere considerata pienamente superata e l'attenzione deve essere ancora alta. in questa fase dobbiamo ripartire e per farlo il Governo e la maggioranza stanno portando avanti tutta una serie di provvedimenti innovativi e necessari. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge semplificazioni rappresenta uno di questi e ci tengo a sottolinearlo. È stato oggetto di un grande lavoro da parte delle Commissioni 1a e 8a, con l'ascolto, l'esame degli emendamenti e riunioni fiume per migliorare un testo accogliendo le proposte migliorative da qualunque parte esse provenissero. Siamo consapevoli che questo provvedimento non è completamente risolutivo rispetto a tutti i problemi legati alla burocrazia, perché un solo testo non può affrontare la cosiddetta giungla normativa prodotta in decenni di leggi, articoli e commi che hanno regolamentato

numerose questioni e in questa fase di ripartenza può dare slancio a settori quali quello dell'edilizia e concretezza ad altri interventi posti in essere dal Governo. Penso, ad esempio, al *superbonus* del 110 per cento sugli interventi di efficientamento energetico per le abitazioni e di prevenzione antisismica. Replicare agli interventi di ognuno di voi richiederebbe ore, ora però permettetemi di soffermarmi su quelli che, anche all'esterno di quest'Aula, hanno maggiormente alimentato il dibattito degli ultimi giorni, non senza letture fuorvianti e strumentali, riprese anche da alcuni interventi in discussione generale. Sulla ricalibratura della responsabilità erariale qualcuno ha ventilato un colpo di spugna. Si è detto che anche la Corte dei conti in audizione ha comunicato che non è opportuno limitare la responsabilità erariale al solo caso di dolo per i funzionari pubblici che firmano la pratica. Abbiamo ovviamente ascoltato con grande attenzione il giudizio della Corte dei conti, ma siamo convinti della bontà della soluzione trovata per superare il contrasto giurisprudenziale e dottrinale e l'atavico problema italiano della paralisi della firma; problema, peraltro, evidenziato in altre occasioni dalla stessa Corte dei conti e da altre autorità indipendenti. Sottolineo, quindi, che non si è fatta alcuna marcia indietro sulla responsabilità erariale, che resta per colpa grave e dolo solo nel caso di comportamenti omissivi del funzionario pubblico a cui è sottoposta la pratica, e la stessa responsabilità viene limitata al solo dolo nel caso del funzionario che firma e che quindi resta perseguibile. Un argomento che, invece, sembra essere sfuggito alle polemiche, ma che vorrei portare all'attenzione anche di chi ci ascolta, riguarda la digitalizzazione. Sul punto possiamo dire che con il decreto-legge semplificazioni è arrivata la svolta. In questo provvedimento c'è la pubblica amministrazione che vogliamo, quella che mette al centro la persona, snellendo le procedure e avvicinando i servizi pubblici ai bisogni e alle esigenze di tutti noi. Rafforziamo il principio del *once only*, un principio vigente da tempo nel nostro ordinamento, ma ancora inapplicato. Le pubbliche amministrazioni non devono più chiedere ai cittadini e alle imprese dati e documenti che già possiedono e che possono reperire da altre pubbliche amministrazioni. Per questo, arriva la piattaforma digitale nazionale dei dati, che deve rendere interrogabili, disponibili e fruibili alla pubblica amministrazione i dati pubblici e conoscibili. Vogliamo poi garantire a tutti gli italiani la cittadinanza digitale e la possibilità del domicilio digitale: tutti i servizi pubblici digitali devono diventare accessibili dal telefono attraverso l'*app* IO, all'interno della quale ciascuno di noi potrà dotarsi degli strumenti di cittadinanza digitale, visualizzando avvisi, comunicazioni e accedendo a tutti gli atti e procedimenti che lo riguardano. Ci sarà anche la possibilità di indicare il proprio domicilio digitale direttamente dall'*app* e i cittadini accederanno a tutti i servizi della pubblica amministrazione con SPID e carta d'identità elettronica. Proprio in questi giorni la ministra Pisano ha annunciato il raggiungimento di quota 10 milioni di SPID attivati. Con il decreto-legge arriva la piattaforma digitale unica per le notifiche di atti e provvedimenti della pubblica amministrazione a cittadini e imprese. La raccomandata cartacea viene sostituita da una comunicazione digitale, ma naturalmente rimane per chi avrà transitoriamente ancora ancora difficoltà con gli strumenti tecnologici. In buona sostanza, quella digitale diventa la modalità normale con cui gli uffici pubblici interloquiscono con i cittadini. Il decreto-legge semplificazioni supera l'impostazione secondo cui le amministrazioni dovrebbero incentivare l'utilizzo del digitale; attraverso l'amministrazione si deve utilizzare il digitale. le pubbliche amministrazioni possono assumere esperti per la trasformazione digitale e hanno l'obbligo di consentire l'accesso da remoto ai dipendenti. Si introduce il dovere per le amministrazioni di misurare e pubblicare i tempi effettivi delle procedure. Tutti potranno mettere a confronto i tempi di attesa. stabiliamo che il ritardo si paga: diversi provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione dopo la scadenza dei termini saranno inefficaci, tranne in caso di atto illegittimo. Presidente, colleghi, non c'è rilancio senza semplificazione. Il nucleo centrale del decreto semplificazioni è costituito da sburocratizzazione, snellimento delle procedure e, come detto, digitalizzazione. Non riusciremmo a cogliere l'importanza di questo provvedimento se non guardassimo ai 209 miliardi per investimenti in arrivo con il *recovery fund.* Si tratta del piano di investimenti più ingente che l'Italia abbia mai visto, ottenuto grazie all'impegno in Europa del presidente Conte. Per questo occorre essere in grado di spendere proficuamente e tempestivamente queste risorse e il decreto semplificazioni darà un grande impulso in tale direzione. Prima di concludere, signor Presidente, mi lasci ringraziare ancora una volta i colleghi di maggioranza e opposizione delle Commissioni 1a e 8a per il lavoro incessante di queste settimane, i membri del Governo la cui presenza costante ha reso proficuo il dibattito parlamentare, gli uffici delle rispettive Commissioni per il loro lavoro indispensabile e quanti, a vario titolo, hanno contribuito a rendere migliore la conversione in legge di questo - a mio avviso - importante provvedimento.

di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, che recepisce sostanzialmente, con alcune correzioni tecniche, le proposte emendative approvate dalla Commissione, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia. Avverto che il testo reca l'inserimento di una ulteriore disposizione particolarmente urgente, volta esclusivamente a prorogare al 30 novembre 2020 il termine per la concessione dei contributi relativi ai danni lievi riportati a seguito del sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016, in scadenza il 20 settembre prossimo. Onorevoli colleghi, la Presidenza ha valutato con attenzione, in costante raccordo con i Presidenti delle Commissioni permanenti 1a e 8a, gli emendamenti presentati al provvedimento in esame. Pertanto, in conformità a quanto già stabilito durante l'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma primo, del Regolamento, tutti Con riferimento agli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite, la Presidenza dichiara, altresì, improponibile, ai sensi della medesima norma regolamentare,

in quanto estraneo all'oggetto del decreto-legge. Conseguentemente, la Presidenza dispone, ai sensi dell'articolo 161, lo stralcio della disposizione identica all'emendamento 19.0.76, contenuta nell'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione presentato dal Governo.

sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1883, di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nel testo dichiarato ammissibile dalla Presidenza. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, trasmette il testo dell'emendamento alla Commissione bilancio, che è fin d'ora autorizzata a convocarsi. Convoco la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il dibattito sulla questione di fiducia. La seduta è sospesa.

quindi sostanzialmente un provvedimento necessario per favorire la ripresa economica del nostro Paese. Si tratta del quarto intervento di questa natura, dopo quelli che abbiamo visto nel passato,

Quando si affrontano temi di questa natura, che hanno impegnato la Commissione fino a tarda notte in più occasioni, credo serva porsi una domanda:

sì. Riteniamo che nel testo ci siano gli strumenti principali per far ripartire l'economia del Paese e per far recuperare e crescere il PIL che è stato perso.

ancora fermi, previsti in più leggi di bilancio, ma che, per varie ragioni, non hanno avuto la loro conclusione. Questo è il motivo fondamentale. Il decreto-legge semplificazioni

possibili, che negli anni sono rimasti fermi nei cassetti, utilizzando le norme di favore del provvedimento. Si tratta di iniziative economiche per diversi miliardi di euro.

mesi, quindi, una svolta epocale. Speriamo che l'Italia sia pronta. Serve uno sforzo, da parte nostra, incentivante rispetto a tutta la macchina pubblica, a sostegno delle istituzioni pubbliche, affinché questo ingente volume di denaro possa dispiegare positivamente i propri effetti sull'economia e quindi a favore della crescita. Molte altre scelte contenute nel decreto-legge incideranno sulla vita reale del Paese. Ho parlato, in particolare, delle infrastrutture, ma contiene anche norme sull'agricoltura, sull'ambiente e sulle innovazioni, tutte decisioni che hanno il merito di snellire e favorire l'attuazione delle delle iniziative in un'ottica positiva, per rendere sempre più tempestivi gli interventi dell'Italia a sostegno, appunto, della crescita. Sono convinto che siamo riusciti a trovare anche quel difficile equilibrio che è sempre difficile da raggiungere - ma credo che ci siamo riusciti e lo sforzo è stato positivo - tra la necessità di crescere e quella di preservare la qualità della vita. Il decreto semplificazioni, quindi, complessivamente è un mezzo utile a disposizione della macchina pubblica. Per questo riteniamo che la sua completa attuazione sia necessaria e, per quanto ci riguarda, doverosa. Valutiamo pertanto positivamente ogni iniziativa a sostegno dell'approvazione

Signor Presidente, è stato svolto un lavoro prezioso e puntuale nelle Commissioni lavori pubblici e affari costituzionali riunite per l'esame del decreto semplificazioni, con l'obiettivo di migliorarlo. Voglio ringraziare i relatori per l'ottimo lavoro svolto, i Presidenti delle due Commissioni e tutti i colleghi commissari per lo spirito di collaborazione manifestato durante i lavori, nel solo interesse di velocizzare il processo burocratico del nostro Paese e di incentivare gli investimenti pubblici durante questo periodo emergenziale. Un lavoro ottimamente mediato dai sottosegretari di Governo Malpezzi e Margiotta, ai quali va il mio personale ringraziamento, e che mi ha arricchito molto per l'importanza dei temi trattati e per il loro elevato impatto sulla vita di tutti i cittadini. Se parliamo di snellimento di procedure, non si può non fare riferimento al tema degli appalti pubblici e degli affidamenti e a quello dei poteri straordinari posti in capo alle stazioni appaltanti per lo svolgimento di lavori sopra soglia e sotto soglia

che rispondono a determinati requisiti, come l'elevato grado di complessità progettuale ed esecutiva e l'impatto che hanno sul tessuto economico e sociale del territorio nazionale, regionale ma anche locale. individuazione dovrà avvenire entro il 30 dicembre del 2020 e per la loro realizzazione o il loro completamento verranno successivamente nominati commissari straordinari. Ma non basta, perché nei successivi sei mesi, quindi entro il 30 giugno 2021, potranno essere individuate altre opere che rispondano agli stessi requisiti appena esposti, alle quali verranno attribuiti altri commissari. Tutto ciò naturalmente sarà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi con tempistiche più ristrette. Insomma, si sta dando seguito a una visione già prevista dal decreto sblocca cantieri e che, ad esempio, ha portato all'individuazione di un'opera strategica per l'Abruzzo e gli abruzzesi: mi riferisco alla messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, un sistema idrico che continui a garantire l'approvvigionamento di acque potabili potabili destinate a circa 700.000 utenti e che, allo stesso tempo, incide sulla sicurezza infrastrutturale e la continuità di funzionamento di una galleria autostradale che attraversa l'Appennino per 10 il traforo del Gran Sasso. Con l'approvazione di un emendamento, abbiamo dotato il commissario straordinario di maggiori poteri, affinché alcune peculiarità particolarmente problematiche che gravitano intorno a quest'opera anche in ambito di dissesto idrogeologico possano essere superate e venga immediatamente dato il via ai lavori. Inoltre, sempre grazie all'approvazione di un emendamento, introduciamo importantissime novità riguardanti il codice della strada. Questo Governo da mesi lavora per favorire il passaggio ad una mobilità più sostenibile e quindi siamo e quindi siamo intervenuti per regolare il traffico in crescita dei velocipedi. Nel codice della strada avremo zone scolastiche dove viene garantita una particolare attenzione ai pedoni e le strade urbane ciclabili che, insieme alle corsie ciclabili, daranno un giusto spazio ai vari velocipedi e sulle quali si potrà viaggiare in piena sicurezza e secondo regole ben definite. In chiusura del mio intervento, voglio soffermarmi sulla tutela garantita per gli usi civici, ottenuta tramite una modifica emendativa al testo del decreto-legge. Infatti, per la realizzazione di opere interrate su terreni che godono di diritto di uso civico, resta la tutela del proprietario allo svolgimento di un *iter* classico - già previsto e in vigore - per la concessione di servitù, sia esso un soggetto privato o un ente pubblico. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il voto di fiducia al decreto-legge semplificazioni diamo una nuova occasione al nostro Paese in questo periodo particolarmente caratterizzato da grandi aspettative nutrite dai cittadini nei confronti

Per essere il «Governo del cambiamento», devo dire che indubbiamente è un bel risultato: cambiamento nel senso di cambiare idea ogni giorno e che

nata e pensata per contrastare la prassi dell'ostruzionismo parlamentare, con ore e ore perse a discutere su migliaia di emendamenti aventi l'unico vero scopo di contrastare l'azione di governo da parte dell'opposizione. Oggi tale procedura è divenuta invece uno strumento

Credo che a tutto ci sia un limite e che il senso del pudore, se non altro, e il decoro delle istituzioni non stiano solo nel venire in Senato Il decoro delle istituzioni attiene - e lo dico alla Presidenza - anche alla possibilità di assolvere a un minimo delle

assurda, alla quale sembra che nessun osservatore voglia prestare attenzione, come ogni cattiva abitudine. Mi veniva in mente questa mattina un parallelo con la falsa fatturazione:

della legalità e della costituzionalità: è prevista in modo specifico in casi assolutamente straordinari, eccezionali e irripetibili. È diventata la prassi assolutamente consolidata di questo Governo: 23 voti di fiducia (questo è il ventiquattresimo) e un solo provvedimento approvato in procedura ordinaria nel nel Conte-*bis*. Tutto ciò da una maggioranza che vede messi insieme i campioni dell'onestà e del cambiamento (anzi, i fenomeni dell'onestà e del cambiamento) e un partito che attinge alla storia repubblicana di anni

confrontarci. Non si può continuare in questo modo. Mi chiedo come sia possibile che l'Istituzione principale del Paese non obietti qualcosa rispetto a questa prassi che è diventata assolutamente consolidata: un ramo del Parlamento resta assolutamente escluso

non per strapparmi i capelli (che sono anche pochi), ma per far presente, colleghi, che a tutto c'è un limite e che anche il decoro delle istituzioni è in capo a tutti noi, in primo luogo alla Presidenza, evidentemente, ma *pro quota*

che non ci ispirate alcuna fiducia. L'impegno della Lega sul provvedimento in esame è stato massimo, nel rispetto del popolo italiano, nonostante il Governo abbia di fatto paralizzato questo Parlamento, riducendo la discussione su un decreto-legge a pochi giorni. Con tale mossa ci sta portando di fatto a un monocameralismo imperfetto, che in realtà è quello che viviamo ogni giorno con questo Governo. Governo. Governo che poi si sta sempre più caratterizzando come autoreferenziale e autoritario: va avanti a colpi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (qui ne abbiamo discussi

annunci roboanti in quest'Aula, promesse senza riscontro, stati generali convocati e conclusi senza un programma ed entità assolutamente misteriose, come le *task force*. Dall'altra parte, c'è la realtà che viviamo sui territori ogni giorno: gli italiani, la vita quotidiana delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese, dei giovani e degli anziani. Il Governo non dimostra alcuna percezione della realtà; ha una sua visione, che racconta un Paese che non esiste, che è in emergenza non da oggi, ma da alcuni mesi da molto tempo ormai); un'Italia in cui la cassa integrazione non è ancora arrivata a tutti, in cui le banche non concedono alle imprese i crediti agevolati e il sistema INPS (il famigerato sistema INPS) va in *tilt* esattamente quando serve, perché quando non serve non va affatto in *tilt*; un Paese in cui gli imprenditori sono spinti più a chiudere che ad aprire. Ricordo che il decreto semplificazioni nasce per adottare misure snelle, veloci ed efficaci, al fine di provare a far uscire l'Italia dalla crisi economica drammatica scatenatasi *post* pandemia; una crisi di domanda e di offerta, per effetto della quale - le previsioni sono di Istat e della Banca d'Italia, non di noi, pericolosi sovranisti - l'Italia uscirà l'Italia uscirà peggio di tutti gli altri Paesi europei, con un crollo del PIL di oltre il 12,4 per cento, una ripresa stimata ai minimi storici per il prossimo anno e una recessione che è quasi il doppio di quella tedesca.

e il 34 per cento ha difficoltà con i pagamenti delle rate e oltre un terzo delle famiglie dispone di risorse finanziarie sufficienti per meno di tre mesi. Si stima che il Paese perderà oltre 800.000 posti di lavoro entro fine anno: una catastrofe. Occorre risolvere i problemi di questo Paese, totalmente abbandonato da un Governo che ha scelto, proprio con questo decreto-legge, di lasciare fuori emendamenti vitali, che avrebbero consentito subito l'impiego degli italiani: quelli per il settore dell'agricoltura,

ci sono 45 milioni di ettolitri di vino da produrre e 25.000 di posti di lavoro per la raccolta delle uve. La difficoltà è enorme. Tutta questa semplificazione che ci ha spiegato il ministro Bellanova non esiste, nemmeno

connesse alla verifica dell'integrità dei serbatoi del GPL, con tempistiche coerenti con l'attuale fase di emergenza e con la possibilità di utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. Abbiamo introdotto anche un reale snellimento delle procedure previste dal codice della strada. Il nostro impegno è stato anche quello di attivarci su emendamenti importanti,

ma particolarmente sentito a livello nazionale. Nel confronto europeo emerge un quadro piuttosto sconfortante per quanto riguarda l'incidenza delle imprese condotte dai giovani. In Italia i giovani con meno di quarant'anni a capo di un'azienda agricola risultano essere l'8 del totale, dato che si pone al di sotto di tre punti percentuali della media europea. Soprattutto, il dato che colpisce è il tasso di ricambio generazionale: mentre in Europa ogni cento capi azienda anziani,

decine di migliaia chiudono, perché non c'è la logica del ricambio generazionale. Ci vogliono investimenti. Magari si parte anche con l'agricoltura 4.0; i giovani vogliono qualcosa di più da questo settore: bisogna aiutarli, ma il ricambio non si fa a parole;

Presidente, un altro tema che mi sta particolarmente a cuore è relativo alla sicurezza sul lavoro e agli infortuni anche mortali come quello che è avvenuto ieri a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, dove Davide Gennero, ventidue

Alla stimata famiglia Gennero va naturalmente la vicinanza dell'Assemblea del Senato e una preghiera, con tanto tanto affetto. Queste sono definite morti bianche ma sono tragedie inaccettabili per un Paese civile, o che perlomeno si definisce tale. Le morti bianche sono tragedie sottostimate dai dati ufficiali. Ebbene, occorre intervenire subito. Occorre investire risorse perché perché non servono solo i controlli, ma serve un'attività di prevenzione verso le piccole e medie imprese che a volte hanno difficoltà ad investire in questo settore. Ricordiamocelo da subito nei prossimi provvedimenti. In conclusione, Presidente, noi non ci fermiamo, non ci arrendiamo. Come Lega non retrocediamo di un centimetro. È vergognoso, e lo dico ora in quest'Aula, il processo contro il nostro *leader* Matteo Salvini, un processo farsa. In realtà vorrebbero processare tutti noi italiani che abbiamo a cuore il nostro Paese. Noi siamo orgogliosi del nostro segretario federale che coraggiosamente ha scelto di difendere l'Italia e gli italiani in tempi non sospetti. Solo nel passato mese di luglio, gli sbarchi sono stati sei volte quelli dello stesso periodo di un anno fa, con la Lega al Governo e con l'arrivo - lo ricordo - di molti clandestini positivi al Covid. L'uso strumentale che voi fate dei *media*, i vostri tentativi di intimorirci e zittirci non ci fermeranno. *(Applausi)*. Come dicevo all'inizio, noi non ci fidiamo e come noi di questo Governo non si fida il popolo italiano. Presidente, processateci tutti! Noi siamo il Paese. Prima gli italiani sempre!

dopo giorni di confronti serrati e discussioni sulla semplificazione di varie procedure irretite da una burocrazia tecnica e su ciò che invece avrebbe bisogno di riforme strutturali e non può chiaramente rientrare in un decreto di emergenza, siamo arrivati ad un testo formulato dal Governo che tiene conto delle misure discusse nelle Commissioni e per cui oggi ci viene richiesta la fiducia. Una fiducia al Governo che reputiamo sia una garanzia per gli italiani italiani che possono contare sulla stabilità necessaria in questo particolare e difficile momento aggravato dalla pandemia non ancora completamente sconfitta. sconfitta. Quello che ci apprestiamo a convertire in legge è un decreto che introduce nel settore dei contratti pubblici e dell'edilizia misure di semplificazione e di innovazione digitale volte proprio ad alleggerire i procedimenti amministrativi pedanti che troppo spesso hanno impedito al nostro Paese di guardare avanti nei settori

tra gli enti, come è avvenuto nell'ambito del procedimento di VIA, con l'esclusione della valutazione ambientale strategica per i piani di sviluppo aeroportuali, così come accade da sempre per i porti. Si interviene anche in altri campi, come nella pubblica amministrazione, con misure che favoriscono l'uso da parte di lavoratori di dispositivi elettronici, personali o messi a disposizione dall'amministrazione stessa, per ottimizzare la prestazione lavorativa e, soprattutto, per fornire migliori servizi all'utenza, senza mai venir meno alla garanzia della sicurezza e della protezione dei dati e delle informazioni a disposizione. Quindi, una agevolazione del cosiddetto lavoro agile. È ovvio che, per realizzare una vera innovazione, come ho detto anche ieri nel mio intervento, sarà necessaria una formazione continua ad ogni livello di servizio della pubblica amministrazione. Formazione continua che deve essere ben strutturata e non può essere delegata

vada ad agevolare i livelli occupazionali, riconoscendo, sempre e in ogni caso, le competenze e il merito di ognuno. Un passo in avanti con questa normativa è stato fatto prevedendo anche la sperimentazione da parte di università, enti di ricerca e società anche per i privati, ampliando così le opportunità per tutti i soggetti che operano in questo campo, senza la limitazione solo ai soggetti pubblici. Soprattutto nei settori della ricerca, si devono democraticamente consentire le stesse opportunità a tutti, soprattutto ai nostri tanti giovani che spesso sono costretti ad andar via dall'Italia. quindi, questo, sia nel pubblico che nel privato, senza preclusioni ideologiche e senza lasciare la gestione miope che c'è stata fino adesso in ambienti che dovrebbero fare cultura e, invece, sono prettamente autoreferenziali. Sono soddisfatta di aver messo fine, e per questo ringrazio il Governo, decreto-legge n. 35 del 2019 (il cosiddetto decreto Calabria) sulla sanità, che aveva causato il blocco delle competenze della stazione unica appaltante regionale, delegando il tutto a convenzioni con altre Regioni, senza espletare alcuna gara e, quindi, senza portare nulla di nuovo alla sanità calabrese, se non consentire una proroga di gare scadute e un aumento di costi per i calabresi. Un interesse preminente è stato dato anche, da parte degli enti territoriali e delle imprese, all'articolo 10 recante semplificazioni ed altre misure in materia edilizia, con cui si introducono le deroghe limiti determinati dalle leggi in questo settore, anche ampliando le definizioni di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia. In fondo, tante modifiche di questo provvedimento, rientrano nell'attuazione del piano *shock* di Italia Viva sulle infrastrutture, presentato al Governo e - sembra - anche condiviso in parte. Considerando il momento di fragilità del nostro Paese, è importante avere tutti l'obiettivo comune di raggiungere gli scopi, anche per le strade più impervie. Solo con il buon governo del Paese può emergere la nostra attività, quella che svolgiamo con serietà e responsabilità, per dare di nuovo senso al ruolo alto e prestigioso delle istituzioni che rappresentiamo.

e, come *extrema ratio*, sulla valutazione penale dei comportamenti individuali. In questi anni, invece, abbiamo avuto un'esponenziale crescita del controllo penale e un'eliminazione dei controlli amministrativi. Il controllo amministrativo non è basato sulla filosofia dell'autorizzazione; la filosofia di una serie di provvedimenti, assunti in particolare nella prima Repubblica, che hanno condizionato la vita dei cittadini sotto il profilo delle libertà.

Si trattava di individuare un elemento scriminante dal momento che quella norma di reato prevede genericamente alcuni comportamenti che sono già determinati da altri reati. reati. La riforma adottata prevede che non ci debba essere discrezionalità nella valutazione. Ci rendiamo conto che, quindi, sarà sempre necessario l'intervento del giudice per stabilire se c'era o meno discrezionalità?

che essa, non solo costringe l'opposizione a votare contro, ma anche a tenere conto della realtà e, cioè, che voi avete impedito un effettivo confronto,

chiunque. Bastava semplicemente avere la capacità di individuare quegli spazi di libertà che dovevano essere riconquistati e dare la possibilità a tutti di intervenire secondo un modello di controllo successivo. (*Applausi*).

Signor Presidente, gentili senatrici e senatori, la fiducia che ci apprestiamo a conferire al Governo questa volta è anche meritata, in modo particolare, da due donne: il ministro per la pubblica amministrazione Dadone e il ministro per l'innovazione digitale Pisano, che, con la loro determinazione, hanno messo in campo delle norme che segneranno la trasformazione digitale del Paese e - sono sicura - ci vedranno già dal prossimo anno fare un significativo balzo in avanti in merito al livello di digitalizzazione del nostro Paese, che verrà immediatamente registrato nell'indice di Voglio elencare brevemente tre delle fondamentali novità in tema di digitalizzazione introdotte dal decreto-legge di cui tutti noi già da subito possiamo beneficiare. Prima però vorrei fare solo un breve inciso per evidenziare come tra gli emendamenti approvati a mia prima firma, oltre a semplificazioni nell'ambito delle procedure di identificazione di acquirenti SIM, dell'Internet delle cose e nell'utilizzo di tecnologie LPWAN, che consentiranno ai cittadini di godere di innumerevoli benefici in termini di digitalizzazione dei servizi e di qualità della vita, vi sia un'importante norma che riguarda il sisma 2012, che ha colpito prevalentemente la mia Regione, l'Emilia-Romagna, finalmente il proseguimento dei lavori di ricostruzione per circa 300 imprese agricole e agroindustriali, che hanno subito gravi danni a causa di questi tragici eventi. Questo Parlamento e questo Governo non si sono dimenticati di voi, agricoltori dell'Emilia-Romagna. Tornando al testo del decreto-legge, al capo 1 del titolo III abbiamo la cittadinanza digitale e l'accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione. È di ieri la notizia che sono state attivate 10 milioni di identità SPID; 10 milioni di cittadini sono pronti ad utilizzare i servizi digitali della pubblica amministrazione. Il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, tramite PagoPA, mette a disposizione il punto di accesso telematico che, dal punto di vista del cittadino, si concretizza nell'app IO. Grazie all'app IO e all'autenticazione che può avvenire indifferentemente con SPID o la con la carta d'identità elettronica, il cittadino può interagire con la pubblica amministrazione centrale e locale in modo semplice, intuitivo, efficace e veloce. Per moltissimi servizi riceveremo una notifica sul nostro *smartphone* e con un semplice clic avremo risolto il nostro problema. L'abbiamo vista in opera con il *bonus* vacanze, la vedremo in azione per pagare il bollo auto, la mensa o lo scuolabus per i nostri figli, per rinnovare la patente o la carta d'identità, per pagare la Tari e progressivamente per tutti i servizi. La notifica ci arriva sullo *smartphone* invece che nella cassetta della posta e la nostra risposta si esegue con un clic. Niente più uffici, sportelli o code, nessun tempo perso. Al fine di garantire la cittadinanza con un clic*,* nel decreto si obbliga quindi la pubblica amministrazione a fornire i propri servizi anche tramite l'app IO e le amministrazioni devono avviare i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.

potrebbero essere lasciati indietro. Infatti per questi piccoli Comuni la data di avvio della trasformazione digitale coinciderà con la fine dello stato di emergenza che stiamo vivendo. Per i loro cittadini il divario digitale sarà quindi acuito. I cittadini dei piccoli Comuni potranno ringraziare la Lega che ha contrattato fino all'ultimo per ottenere di creare questi cittadini digitali di serie B

Questo è un forte incentivo a non introdurre ritardi, che andrebbero solo a penalizzare i cittadini e il loro diritto alla cittadinanza digitale. Il decreto, al capo II del titolo III, introduce delle norme in materia di sicurezza nazionale cibernetica. Il testo della norma si preoccupa di diffondere la modalità di lavoro agile contestualmente all'adozione di ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli *standard* nazionali europei e internazionali per la protezione delle proprie reti. Si promuove la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei dispositivi attraverso apposite linee guida, con particolare attenzione ai servizi erogati tramite fornitori di servizi *cloud*. Tutti i servizi informatici della pubblica amministrazione, in particolar modo quelli *in cloud*, dovranno attenersi al codice di condotta tecnologica, che regola le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. La sicurezza dei nostri dati sarà quindi al centro dell'attenzione, della progettazione e della gestione dei servizi digitali. Nel capo III si sancisce la strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali, mediante la disponibilità e l'interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, oltre ad alcune semplificazioni per la piattaforma digitale nazionale dati. L'obiettivo è che finalmente le banche dati possano colloquiare l'una con l'altra, in modo tale che finalmente possa essere operativo il principio *once-only*. La pubblica amministrazione non può più chiedere al cittadino informazioni, che già le sono state conferite e che la pubblica amministrazione conosce già: ciò comporterà un notevole risparmio di tempo per tutti e una notevole riduzione degli errori, che involontariamente si compiono ogni qualvolta i dati transitano nelle mani di operatori umani. Giungiamo infine al consolidamento e alla razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese: il famigerato *cloud* della Tutti noi abbiamo interiorizzato il concetto di sovranità digitale e questo è sicuramente il nostro obiettivo, perché da questa sovranità derivano i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini del presente e del futuro. Il principio della sovranità digitale è un obiettivo da raggiungere per tutta l'Europa e che attualmente l'Europa non ha

L'unica prospettiva per questo recupero è che avvenga per tutta l'Europa insieme. L'Italia sicuramente non può fare da sola. La prospettiva di *cloud* della pubblica amministrazione, presentata dall'articolo 35 del decreto-legge, si inserisce in una strategia a lungo termine, di cui questo è solo il primo passo, ossia il consolidamento dei servizi. Non possiamo più permetterci la farraginosità di 11.000 *data center* energivori a insicuri. Per questo primo passo potremmo usare i poli strategici nazionali oppure il *cloud* pubblico, differenziando oculatamente la collocazione dei servizi e applicando scrupolosamente il codice di condotta tecnologico. Contemporaneamente dovremo far progredire e crescere le nostre aziende nazionali, che hanno il loro *business* nella fornitura di infrastrutture per il *cloud* e nello sviluppo di servizi applicativi e di *software*. Teniamo presente che, nei prossimi cinque anni, il valore dell'economia dei dati, in Europa, passerà dagli attuali 300 miliardi di euro ad 830 miliardi di euro, con una crescita del 2,4 per cento del PIL totale europeo. Il digitale è l'unico settore che prospetta queste *performance*, ma l'Italia ne potrà beneficiare? Solo se avremo i professionisti che si dedicheranno a queste attività, in particolare i programmatori di *software*. Oggi in Europa abbiamo 5,5 milioni di questi professionisti e nel 2025 avremo bisogno del doppio,

Per questo tutti i Paesi vanno alla ricerca di queste professionalità, anche formate negli altri Paesi, per accaparrarseli. Quindi, il nostro problema da una parte è formare le professionalità per far sviluppare il nostro Paese e nello stesso tempo riuscire a trattenerle, per non farle migrare. La sfida di *next* *generation* EU è soprattutto ovvero quella di riconvertire una buona fetta della forza lavoro in professionalità informatiche di alto livello e di impiegarle per la modernizzazione del Paese e per la gestione della sicurezza dei dati dei nostri cittadini. In questo investimento sta il segreto della crescita e della prosperità del nostro Paese e, nel contempo, della libertà e dei diritti di tutti i nostri cittadini. I nostri Ministri lo hanno capito e hanno iniziato questo progetto: noi sicuramente le sosteniamo e convintamente sosteniamo gli obiettivi di questo decreto.

onorevoli colleghi, in relazione all'andamento dei lavori della Commissione bilancio sul maxiemendamento, sentito il Presidente del Senato, sospendo nuovamente la seduta.

Signor Presidente, visto che c'è stata un'interlocuzione da parte di tutti i Capigruppo per cercare di sveltire la procedura, volevamo ringraziarla per la cortese attenzione che ha avuto nei nostri confronti nell'accordarci la possibilità di iniziare le dichiarazioni di voto, perché comunque da parte di tutti c'era la volontà di mantenere

anche quelli di noi che sono abituati a fare politica come si faceva una volta, in mezzo alla gente, si devono rassegnare. Viviamo nell'era della comunicazione e questa maggioranza lo ha capito bene lo ha capito bene perché conosce le regole. Sa che le parole hanno sicuramente una grande importanza nel mondo della comunicazione attuale. È per questo che gli italiani hanno dovuto sorbirsi una serie di proclami belligeranti, una serie di trasposizioni della realtà che poi, alla fine, non hanno avuto i contenuti che tutti speravamo. Abbiamo sentito parlare di cura Italia, di decreto liquidità, di decreto rilancio, il tutto condito da quello che Conte ha voluto mettere in campo rilanciando - questa volta il termine va usato - le famose parole «potenza di fuoco». Abbiamo ascoltato addirittura il Presidente del Consiglio che parlava di potenza di fuoco con la quale sarebbero stati risolti i problemi delle imprese e dei cittadini italiani. Mentre io sto parlando, mentre noi parliamo, centinaia di aziende in Italia ancora non hanno preso i soldi e centinaia, migliaia di lavoratori - quelli più deboli, quelli delle piccole aziende - ancora non prendono la cassa integrazione. Ecco la potenza di fuoco del Governo Conte.

con le parole roboanti. Adesso ci accingiamo a votare, tramite l'ennesimo ricorso alla fiducia, quella che il presidente Conte ha definito la madre di tutte le riforme: il decreto semplificazioni di oggi dovrebbe essere, secondo Conte e secondo questa maggioranza, la madre di tutte le riforme. Certo che la parola ci sta tutta, una parola evocativa, una parola magica, perché ogni cittadino italiano, ogni impresa ha dovuto duellare con la burocrazia in Italia,

un provvedimento che interviene in maniera disorganica e disarticolata in diversi ambiti e che assume i connotati di un decreto *omnibus*, una summa nella quale si trova tutto e il contrario di tutto, dalla disciplina sui contratti pubblici al diritto di voto per gli italiani all'estero, passando per l'abuso d'ufficio, all'identità digitale, i porti, i viadotti, le università, l'Alitalia, la valutazione sull'impatto ambientale; materia quest'ultima che mi è molto cara perché, con grande delusione, ho visto bocciare i miei emendamenti sui siti di interesse nazionale, relativamente alle decine di migliaia di aziende che stanno delocalizzando perché in Italia non è possibile, per chi ricade nei SIN, spostare nemmeno un cancello. Con le associazioni di categoria, con le associazioni ambientaliste e con i Comuni

bocciati, sacrificati sull'altare di una semplificazione che non semplifica nulla. Per questo sono costretto a dire, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, che l'unica semplificazione che avete fatto e che avete ottenuto è quella delle procedure parlamentari, perché state mortificando la nostra azione politica, la nostra rappresentanza e questo Parlamento

Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, oggi, per Italia Viva è un giorno di festa. Aver portato all'attenzione di questa maggioranza e poi di questo Parlamento quello che abbiamo definito il piano *shock* e che oggi assume la denominazione di decreto semplificazioni è un risultato politico importante. Nel momento in cui diciamo che sbloccare i cantieri serve a far ripartire l'Italia, diamo atto al Governo di essere stato di parola. Un osservatore dei tempi che stiamo vivendo che io ammiro molto, che si chiama Massimo Recalcati, sostiene che c'è un tabù nel dibattito politico di oggi. È il tabù della gratitudine. È come se esprimere gratitudine fosse un qualcosa di talmente fuori moda, *démodé*, inconsueto, da suonare strano. Io qui, oggi, voglio esprimere gratitudine verso il Presidente del Consiglio, verso i membri del Governo, verso la maggioranza, verso tutto l'arco parlamentare, perché oggi si fa chiarezza su un punto che noi di Italia Viva avevamo posto. Quando, lo ricorderete, perché la maggioranza la maggioranza lo ha osservato e l'opposizione ci ha attaccato, noi abbiamo posto un tema di distanza e di dissidio, anche nei confronti della maggioranza, in un determinato momento nella primavera del 2020, molti osservatori hanno detto: chissà cosa chiederanno quelli di Italia Viva, quanti posti, quanti Sottosegretari, quanti Ministeri. Ebbene, i posti sono sempre quelli di prima. Noi non abbiamo chiesto posti, ma abbiamo chiesto l'assunzione della responsabilità politica di dire che questo Paese riparte dalle infrastrutture e dai cantieri, dai sussidi e dall'assistenzialismo. Il Presidente del Consiglio, su questo, è stato di parola, perché il decreto semplificazioni è la risposta alle nostre richieste. È sufficiente? Lo vedremo. Non è l'atto che noi sognavamo, ma riconosciamo che in quell'atto c'è molto di quanto chiedevamo. E riconosciamo che questo è stato possibile per uno sforzo da parte di tutti, ma anche perché dobbiamo imparare dalla storia del nostro Paese. La storia del nostro Paese è una storia nella quale, se guardiamo gli ultimi anni, gli episodi di maggiore successo sono quelli che hanno visto la presenza, come il decreto semplificazioni prevede, di commissari e di procedure semplificate. Astrattamente, questo è discutibile. In un Paese normale, le cose funzionerebbero a prescindere dalle strutture commissariali. Ma chi fa politica affronta la realtà, non il proprio pregiudizio ideologico. Se oggi Pompei non fa più notizia per i crolli, ma fa notizia perché le persone sono tornate a riscoprirne la bellezza, è perché si è scelta una procedura commissariale anno fa, a un importante generale dell'Arma dei carabinieri. Se l'Expo ha permesso a Milano di tornare ad essere una capitale europea, è stato grazie a quelle strutture commissariali che hanno permesso la realizzazione di un evento che, nella primavera del 2014, sembrava impossibile. Allo stesso modo, il ponte di Genova oggi sta lì a dimostrare che l'Italia sa fare le cose per bene se vuole. Accanto a questo, però, signor Presidente, abbiamo il dovere della franchezza. Ci sono delle pagine, anche adesso, di brutta politica. C'è il ponte di Genova che, con il dolore dei caduti e con la capacità degli operai, è ripartito, ma c'è anche un ponte, a pochi chilometri di distanza, al confine tra Liguria e Toscana, il ponte di Albiano Magra, che è caduto, si è accartocciato su se stesso sei mesi fa e che è ancora lì nelle stesse identiche condizioni. Nel momento in cui io dico bravo e ringrazio per aver sbloccato il piano *shock*, io dico anche al Governo che si deve fare molto di più. Non è, infatti, pensabile che quell'episodio, che non ha fatto notizia semplicemente perché, fortunatamente, in pieno *lockdown* non ci stava passando praticamente nessuno, sia un episodio di serie B. Ci sono tanti ponti,

Provo rapidamente a sintetizzare le tre sfide che, secondo me, abbiamo di fronte. La prima è un tema che riguarda le città d'arte. Noi dobbiamo avere consapevolezza che le città d'arte rischiano di essere spazzate via dalla pandemia, almeno nel breve periodo. Certo, nessuno ammazzerà mai Firenze, Venezia o Roma, ma queste città hanno una sofferenza doppia. doppia. In questo decreto sono inserite misure importanti per alcune città. Da senatore eletto nel collegio di Firenze sono molto felice della norma prevista non dai lavori parlamentari, ma direttamente dal Governo sullo sblocco dell'aeroporto e sono molto felice del fatto che si capisca che l'investimento sugli stadi non è un giocattolino per i tifosi,

Lo dico con molta forza: dobbiamo avere l'intelligenza, come ha proposto, ad esempio, un funzionario dello Stato, il prefetto di Firenze, di andare verso il sistema delle zone franche urbane nelle città d'arte - vedo persone che conoscono le città d'arte per tanti motivi - oppure avremo una sofferenza

tra chi crede che la ricostruzione passi dai ponti e chi pensa che la ricostruzione passi dai muri. Non voglio citare il grande pensiero di Giorgio La Pira, ma nel momento in cui si riparte si deve scegliere il modello culturale che si vuole per il Paese. Io penso - lo dico con rispetto verso i compagni di esperienza, ancorché avversari politici, di Fratelli d'Italia e della Lega - che l'idea del sovranismo abbia mostrato i suoi limiti e ne abbiamo già parlato. Penso che il *lockdown* abbia dimostrato come l'Italia abbia tutto tranne che l'esigenza del sovranismo. L'Italia è un Paese che ha bisogno di essere spalancato sul mondo; ha bisogno di globalizzazione e di essere aperto perché, se blocchiamo

temi. Noi abbiamo un'enorme quantità di denari (208 miliardi di euro) che vengono dall'Europa e che devono essere spesi nelle prossime settimane, mesi e anni. Su che modello di sviluppo li mettiamo?

a intervenire cercando di far sì che il coronavirus fosse innanzitutto bloccato. Vorrei che da quest'Assemblea arrivasse un messaggio anche in queste ore di grande vicinanza e affetto per tutti coloro che sono ancora in prima fila a combattere contro il coronavirus, ovvero gli infermieri, i medici e anche chi sta soffrendo per il coronavirus. (*Applausi*). Signor Presidente, per il suo tramite vorrei rivolgere un affettuoso augurio di pronta guarigione al presidente Silvio Berlusconi perché penso che questo sia un segnale di grande rispetto verso un uomo delle Istituzioni del quale sono stato e sono avversario politico, ma che in questo momento sta vivendo un momento di difficoltà. (*Applausi*). Signor Presidente, una volta che abbiamo detto che il coronavirus c'è ed è l'occasione di combattere contro un grande problema, ma anche di ripartire, l'ultimo punto è molto semplice: dopo le elezioni regionali, il Governo e la maggioranza dovranno avere la forza di venire in Parlamento e chiarire in modo organico, strategico e visionario, se possibile, come intendiamo affrontare la grande occasione del *recovery* *fund*, dei 200 miliardi e - io dico - anche del MES e del programma SURE. Mi spiego in un altro modo: dobbiamo venire in Parlamento a spiegare il il nostro disegno per i prossimi tre anni oppure non ci sarà possibilità alcuna per la politica di svolgere un ruolo. Per dico che il Governo, che fortunatamente rispetto al Governo precedente segue più Macron e Merkel che i *gilet* gialli e Alternative für Deutschland, deve prendere esempio da ciò che ha fatto Macron ieri: 100 miliardi, 20 pagine spiegate bene e una visione per i prossimi anni. Dopo le elezioni regionali attendiamo il Presidente del Consiglio in Aula per un grande dibattito su questi temi. Nel frattempo, Italia Viva vota la fiducia convintamente. Il piano *choc* è diventato legge; ha vinto l'Italia, ha vinto la politica.

urgenza, all'insegna del fatto che era necessario sostenere le famiglie, le imprese, garantire la cassa integrazione e il reddito d'emergenza. una serie di provvedimenti che sono stati, a mio avviso, assolutamente fondamentali. Il decreto-legge affronta un'altra questione, che è quella della semplificazione e delle velocizzazioni per la ripresa dei lavori e delle opere, per dare

certamente con le semplificazioni e si è operato con le deroghe, che sono previste nel provvedimento per quanto riguarda tutto il sistema dei contratti pubblici, delle gare e degli appalti. La

di personale qualificato e di tecnici. Per troppo tempo, soprattutto le amministrazioni comunali e gli enti locali, ma anche l'apparato dell'amministrazione centrale, a causa del blocco del *turnover*, sono stati ridotti praticamente all'osso. Noi abbiamo bisogno di investire nelle risorse umane, nei giovani e nella qualificazione del personale. Come è infatti noto i tempi lunghi vengono prima di andare in gara, nella fase della progettazione. Questa è quindi l'altra scommessa che non possiamo assolutamente perdere. Servono investimenti

il ministro Bellanova, che sa bene che nella sua Regione ci sono dei gioielli, anche nei posti più inaspettati, dei centri storici e un tessuto prezioso dal punto di vista edilizio. Su quello sosteniamo che ci vuole cautela. Certamente si devono fare interventi, ma all'interno di un piano di recupero e di riqualificazione, in cui le amministrazioni pubbliche, le amministrazioni comunali, sappiano gestire e indicare qual è il piano di riqualificazione.

anche sociale ed economico enorme, che dobbiamo preservare e migliorare. Questa è stata la portata del lavoro che abbiamo compiuto. Abbiamo affrontato anche altri temi e abbiamo corretto norme: pensiamo alla questione della valutazione di impatto ambientale. Abbiamo restituito tempo alla discussione pubblica e ai cittadini, per poterli coinvolgere, perché la partecipazione alle opere è un fatto fondamentale, affinché i cittadini sappiano e conoscano.

dico subito che voteremo convintamente la fiducia su questo provvedimento, un provvedimento che, com'è stato detto da diversi colleghi che mi hanno preceduto, riteniamo importante per il Paese. un decreto che qualifica l'azione di Governo e che ci consente di affrontare meglio la ripartenza dopo il Covid; un provvedimento che esce arricchito e migliorato dal confronto parlamentare, dal lavoro positivo della maggioranza e dal contributo della stessa opposizione, a cui vorrei dire che non si può, da una parte, sbandierare l'approvazione di decine di propri emendamenti e poi però denunciare la presunta mancanza di volontà

Ancora, voteremo la fiducia su un provvedimento davvero utile al Paese: si può dire e dovremmo dirlo tutti anche perché, al di là delle parole, della propaganda e delle volgarità - anche oggi ho sentito il senatore Salvini dire dire che il Governo è criminale - al di là di tutto questo, appunto al di là della propaganda dell'opposizione, se non fosse un provvedimento molto utile per il Paese, dovreste spiegarci perché avete proposto e ottenuto di prolungarne di cinque mesi gli effetti. Questo provvedimento dimostra che è possibile velocizzare le opere, ridurre i tempi senza rinunciare alle regole, alla trasparenza e alla tutela del lavoro. Si possono ridurre i tempi e i vincoli burocratici senza sospendere - come vorrebbe qualcuno o, meglio, come avrebbe voluto qualcuno - il codice antimafia o il codice degli appalti. Dimostreremo ai teorici del baratto «più opere, se c'è meno legalità» che invece è possibile e giusto tenere insieme le cose. Sulla convinzione che si debbano ridurre i tempi e la burocrazia senza eliminare le tutele di legalità e le regole, il Governo e la maggioranza hanno costruito - io credo bene - questo provvedimento. Questa è la cifra del decreto: liberiamo risorse enormi per appaltare opere pubbliche e infrastrutture, accelerando le gare e non rinunciando alla trasparenza. Inoltre, dopo gli emendamenti che abbiamo proposto e che sono stati approvati sulla pubblicazione dei bandi e sulla rotazione delle aziende per gli appalti sopra soglia, abbiamo ulteriormente migliorato l'aspetto della trasparenza. Anche sull'edilizia ora la collega De Petris - non solo la norma, così com'è uscita dalla discussione di questi giorni, semplifica in modo significativo gli *iter* amministrativi e autorizzativi, ma lo fa senza togliere ai sindaci e agli amministratori le prerogative rispetto alle scelte urbanistiche.

bisogna dire chiaramente che qui ci sono già l'abbattimento e la ricostruzione di edifici esistenti che devono essere sostituiti, che viene considerata una semplice ristrutturazione e non una nuova costruzione. Sarà consentito intervenire sulle sagome e aumentare le volumetrie. Basterà, nella maggioranza dei casi, la semplice segnalazione di inizio attività.

Con un emendamento presentato insieme al senatore Collina abbiamo consentito di realizzare - solo con la SCIA e senza bisogno del permesso di costruire - anche nuove costruzioni di interesse pubblico: scuole, ospedali, edilizia sociale; tutto questo accelera. E non è neppure vero che questo provvedimento blocca gli interventi nei centri storici. Per tali interventi continuerà a servire il permesso a costruire; certo, non potranno essere omologati a semplici ristrutturazioni, ma l'abbattimento e la ricostruzione restano possibili, anche modificando le sagome e le volumetrie, se coerenti con gli strumenti urbanistici comunali e regionali. Sostenere che questo è un provvedimento che serve a impedire l'abbattimento e la ricostruzione di immobili obsoleti è sbagliato; per contro, sostenere che un provvedimento come questo deve anche servire a impedire l'abbattimento e la ricostruzione di immobili di pregio penso sia giusto. Non è vero che è un blocco degli interventi; è semplicemente una scelta per salvaguardare un patrimonio culturale e storico di questo Paese. In realtà, sulla materia edilizia c'è una semplificazione importante che può creare lavoro e migliorare le città, fatta con equilibrio, tenendo insieme necessità di fare presto, tutelando il patrimonio storico, culturale e di pregio. C'è molto altro signor Presidente, che dovrebbe essere valorizzato. Mi limito a tre sottolineature perché i miei colleghi durante il dibattito hanno già affrontato molte questioni. La prima riguarda innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione: una parte importantissima del provvedimento, che renderà concretamente la vita più semplice a famiglie e imprese, mettendo la pubblica amministrazione nelle condizioni di essere più vicina ai cittadini e di dare risposte più rapide a cittadini e imprese. Il secondo elemento che voglio valorizzare è frutto del lavoro dei Gruppi e dell'interlocuzione con i Comuni. Mi riferisco agli emendamenti approvati sulla mobilità nelle città, che danno più strumenti per organizzare la mobilità evitando che il post-Covid, con le difficoltà di utilizzo del trasporto pubblico, ci faccia tornare indietro a un uso diffuso e prioritario dell'automobile, con le conseguenze devastanti che avrebbe su traffico e ambiente. Infine, vorrei dire a chi l'ha sostenuto che non è stato abolito alcun reato. Sull'abuso d'ufficio si è trovato - anche qui - un equilibrio migliore; c'è la necessità di dare maggiori certezze e tranquillità a chi si assume responsabilità nella pubblica amministrazione. Sostenere che se non c'è dolo non può esserci punibilità è giusto, così come ritenere che, se una norma lascia spazi di discrezionalità, il reato eventualmente commesso non può essere l'abuso d'ufficio. Dall'altra parte, è giusto che diventi una responsabilità da sanzionare quella di chi non si assume la responsabilità fino in fondo di garantire tempi congrui ai procedimenti autorizzativi. Questo dice il provvedimento.

Lo voglio dire a tutta la maggioranza: dobbiamo essere orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, di aver scelto la seconda strada, quella della responsabilità e della consapevolezza che, oggi più che mai, il nostro dovere è aiutare famiglie e imprese a ripartire, in un Paese che funzioni meglio. Il provvedimento in discussione

Signor Presidente, esponenti del Governo, colleghi senatori, vorrei preliminarmente, se me lo consentite, visto che sento il dovere di ringraziare il senatore Matteo Renzi per averlo fatto, rivolgere un pensiero affettuoso e accorato al nostro presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Essendo stato ricoverato questa notte presso l'ospedale San Raffaele, a lui, a nome di tutto il Gruppo Forza Italia, rivolgo il più affettuoso augurio che possa tornare tra noi nel più breve tempo

nostro è un movimento politico nato e cresciuto intorno proprio all'idea che questo Paese divenisse più semplice, più facile per i cittadini italiani, quindi parlare di semplificazione per noi significa tutto. Capite bene che per un movimento politico che basa il suo pensiero e la sua azione sul mettere al centro delle proprie attenzioni, del proprio agire politico e non lo Stato, non il pubblico, l'idea di realizzare un provvedimento come questo era di straordinaria importanza e soprattutto di straordinaria portata politica. È questa la ragione per la quale ci eravamo già mossi in precedenza e quando il Presidente del Consiglio dei ministri, a fronte delle nostre proposte e delle nostre richieste anche di abrogazione del codice degli appalti, ha avviato l'idea di realizzare un decreto-legge che si occupasse esattamente di questo compito a largo raggio, parlando non solo di codice degli appalti, ma anche di edilizia privata, privata, di terremoto e di altri temi di grande urgenza ed attualità per il nostro Paese, noi l'abbiamo colta come un'occasione importante. È questa la ragione per la quale noi di Forza Italia ci siamo posti ancora di più in una logica di collaborazione con il Governo e con la maggioranza. Ebbene, devo dirvi che anche in questa occasione, purtroppo, il sentimento che emerge tra noi è la delusione. Noi siamo profondamente delusi. *(Applausi)*. Siamo delusi innanzitutto per un concetto, che evidentemente è nella mente e nel cuore del presidente della Repubblica Mattarella, ma non degli esponenti di questa maggioranza, e cioè che questa pandemia, questa epidemia di *coronavirus* che ha colpito il nostro Paese e non solo, poteva e doveva essere una straordinaria opportunità, una straordinaria occasione per ottenere due risultati: in primo una vera coesione nazionale, un'unità di popolo che mettesse insieme non solo quelli che votano per voi, ma anche quelli che votano per noi, che oggi sembrano essere la maggioranza. Nei momenti di difficoltà, così come è accaduto anche in passato, penso ad esempio al dopoguerra, il popolo deve essere unito se vuole raggiungere alti obiettivi, non può dividersi, e mai come in questa occasione avevamo l'opportunità di farlo. In secondo luogo, quando capitano tragedie di questa portata, portata, vige il principio dell'ora o mai più. *(Applausi)*. Questa poteva essere un'occasione straordinaria per sbloccare il nostro Paese da una terribile cultura del sospetto che da trent'anni blocca ogni attività di questo Paese.

di vera e autentica collaborazione: non abbiamo predisposto emendamenti ostruzionistici, ma abbiamo proposto emendamenti, in particolare quelli che abbiamo segnalato agli esponenti della maggioranza, che volevano portare questa maggioranza a condividerli per sbloccare alcuni problemi che attanagliano il Paese e che vengono sottolineati anche da alcuni esponenti della vostra maggioranza. Poco fa ho ascoltato Matteo Renzi, il quale ha posto come una delle prime emergenze di questo Paese lo sblocco delle opere pubbliche e la realizzazione di infrastrutture. È giusto ricordare che che l'Italia, dopo la Seconda guerra mondiale, ha messo insieme tutte le energie, tutte le risorse e tutto il potenziale di creatività di cui è capace il popolo italiano per rinascere, e nel giro di pochi anni siamo diventati un esempio per gli altri Paesi in Europa. Siamo stati il primo Paese a realizzare un'autostrada in Europa; ma sapete che oggi siamo gli ultimi per opere pubbliche? *(Applausi).* Abbiamo una capacità di realizzare infrastrutture pari a zero; qualunque altro Paese riesce a realizzarle in modo molto più rapido e semplice. Soprattutto, quel che abbiamo realizzato negli anni passati purtroppo sta cadendo a pezzi. Il crollo del ponte di Genova è non solo l'aspetto di una inefficienza di chi gestiva quell'autostrada, ma è un problema che riguarda tutte le opere pubbliche di questo Paese, tutta la rete autostradale, i nostri ponti, le nostre strade, i nostri ospedali, persino i nostri edifici comunali. Noi abbiamo bisogno di far ripartire questo Paese *(Applausi),* perché senza infrastrutture resta piantato, muore.

È un'impostazione ideologica e di mancanza assoluta di fiducia nel popolo italiano - questa è la verità - che purtroppo ha fatto sì che negli ultimi anni questo Paese raggiungesse livelli davvero infimi infimi rispetto agli altri. Siamo divenuti negli anni Ottanta la settima potenza economica mondiale. Signor sottosegretario Margiotta, lo sa che non lo siamo più? Lo sa che ormai siamo stiamo diventando il fanalino di coda? Non riusciamo più a realizzare opere; qualunque cosa riusciamo a bloccarla in tutti i modi possibili e immaginabili. Volete qualche esempio degli emendamenti che voi avete respinto? Abbiamo portato avanti alcuni emendamenti con il chiaro ed evidente con il chiaro ed evidente intendimento di cercare di semplificare la vita agli italiani. L'ha detto poco fa il collega Caliendo: il problema è quello dei controlli esasperati, di tutti i controlli *ex ante*; in questo Paese non è possibile fare i controlli *ex post* perché non siamo in grado di farlo come in tutti gli altri Paesi moderni e anglosassoni? *(Applausi).* Non è possibile. Abbiamo fatto questo tipo di tentativo sperando di trovare un po' di collaborazione, ma purtroppo - diciamocelo francamente - la vostra maggioranza è divisa al suo interno: dentro di voi ci sono culture ambientaliste, giustizialiste, culture del blocco, culture del sospetto, con le quali, purtroppo, vi trovate a dover confliggere quotidianamente. Anche soltanto un intervento quale quello sugli stadi,

Perché ci sono ancora alcune predisposizioni ideologiche che purtroppo bloccano ogni intervento possibile che stimoli il rilancio dell'economia di questo Paese. I migliori giuristi, i migliori i migliori amministrativisti, sanno perfettamente che questa è una condizione unica nella storia di questo Paese ed è l'unica condizione che ci può far trovare pronti per un rilancio dell'economia. questa era una buona iniziativa. Come ho detto all'inizio, il decreto semplificazioni poteva essere un'occasione, un'opportunità unica per rilanciare la nostra economia. solo in parte viene colto questo aspetto. Il codice degli appalti, che fu approvato durante il Governo Renzi, ha purtroppo bloccato ogni iniziativa infrastrutturale;

blocchino tutto attendendo il merito, non dando più alcun tipo di sospensiva e bloccando quindi l'intervento,

è stato sostanzialmente un ostracismo nei confronti di tutte le idee sane che noi abbiamo portato nell'interesse dei cittadini italiani e che non sono state colte. Noi ci auguriamo che, sia pure in modo indiretto, qualche processo di di miglioramento possa comunque emergere da questo provvedimento. Tuttavia, tenuto conto dell'atteggiamento ideologico o *post* ideologico che ancora alberga in questa amministrazione, che non ha dato la possibilità ai nostri migliori contributi di essere approvati per qualificare meglio questo provvedimento, noi saremo costretti ancora una volta a votare no. *(Applausi)*. Il Gruppo Forza Italia voterà contro questo provvedimento.

Il *premier* Conte e la maggioranza, come al loro solito, l'avevano sparata grossa. Avevano promesso - non a noi, ma agli italiani - che con questo provvedimento, dopo la povertà, avrebbero abolito anche la burocrazia. Pur non avendo grande fiducia nelle roboanti dichiarazioni delle conferenze stampa e delle dirette Facebook, ci siamo messi in gioco, perché era comunque un'occasione per dare risposte concrete al Paese. Un'occasione attesa da amministratori locali, associazioni di categoria e imprese. Una richiesta forte, che arriva da tutti i cittadini, è che la normativa con cui ci troviamo ad agire sia certa e non in continuo cambiamento. In pratica, l'aspettativa di un Paese moderno, un Paese del G7, era che le semplificazioni divenissero strutturali, superando il codice degli appalti, che - ormai è evidente a tutti - ha di fatto bloccato gli interventi, le opere infrastrutturali e gli investimenti, e dall'altro facilitando la vita ai cittadini. I nostri emendamenti andavano in questa direzione, ma non avete voluto ascoltare chi dal punto di vista amministrativo ha sicuramente più esperienza di buona parte della vostra maggioranza *(Applausi)*, visto che la maggior parte dei parlamentari dei 5 Stelle non ha mai messo piede in un consiglio comunale e ancor meno nella Giunta di un Comune. Siete passati dal divano e dai vostri *blog* alla guida del Paese, e infatti i risultati si vedono. Non avete voluto considerare la moratoria sul codice degli appalti. Per lo meno siamo riusciti, ma solo dopo un'insistenza da sfinimento, a farvi capire la necessità di prorogare i termini del decreto semplificazioni fino al dicembre 2021. Anche in questo caso siete stati un po' tirchi e soprattutto poco lungimiranti, visto che avevamo chiesto di arrivare fino al 2023. Vogliamo scommettere che diversi dei provvedimenti adottati nel decreto semplificazioni finiranno nel prossimo mille proroghe? Il contrario di quanto ci chiedono i cittadini e le imprese: invece di norme certe, lungimiranti, strutturali, di largo respiro, voi continuate a mettere toppe che però non danno certezze e possibilità di programmazione. Una sperimentazione come questa avrebbe avuto la necessità di un tempo più ampio per capirne gli effetti reali. Siamo dispiaciuti che alcune nostre proposte di buon senso non siano state recepite. Secondo noi alcuni articoli porteranno a svariati contenziosi e intoppi burocratici. Un esempio? La responsabilità del RUP

in cui invece ora vi siete chiusi dentro a chiave, e andaste tra la gente, nei cantieri e nei Comuni, vi rendereste conto che non è il RUP che blocca gli interventi, ma la burocrazia che voi state complicando, anziché semplificando, solo perché si vede malaffare e corrotti in ogni amministratore. *(Applausi)*. Voi così però offendete e umiliate migliaia di sindaci, assessori, consiglieri e dipendenti comunali, che lavorano con impegno e onestà al servizio della propria comunità. Ma voi che siete rimasti chiusi nel palazzo e nei vostri *blog* non potete sapere il mazzo che si fanno realmente nei Comuni. Ancora: quanti contenziosi partiranno sull'esclusione dalla gara di imprese di cui si ha conoscenza di non aver ottemperato a contributi o imposte? È così che pensate la ripresa dell'economia e di aiutare le imprese? Impedendo loro di avere un appalto della presunta conoscenza di non aver versato delle imposte? Magari era meglio ascoltare le nostre proposte per superare questo punto e prevedere la possibilità di accordi di rientro. Non avete voluto capire cosa comporterà il fatto di non aver tolto il riferimento negli atti di trasferimento delle piccole deformità, uno snellimento per le autorizzazioni paesistiche per dare la possibilità a tutti di usufruire del *superbonus* in edilizia. visto il momento difficile che stiamo vivendo, non avete concesso la possibilità di deroga per tutti i porti italiani per interventi infrastrutturali, così come concesso al porto di Taranto. Bisogna sottolineare, però, che diversi nostri emendamenti sono stati accolti e di questo vi diamo atto, perché in questa occasione rispetto ad altri provvedimenti la voce del buon senso è stata ascoltata. *(Applausi)*. Certo, abbiamo dovuto insistere non poco e per questo permettetemi di ringraziare i colleghi della Lega per il lavoro svolto con proposte concrete, fatte di esperienza e ascolto del territorio. Siamo riusciti a far comprendere che erano urgenti le semplificazioni per sbloccare gli appalti per gli enti locali e per i disabili, per risolvere le annose problematiche delle motorizzazioni civili. E ancora, visto l'accumulo di pratiche inevase, la proroga del termine per la restituzione del beneficio fiscale per quelle imprese che dal 2010 al 2012 hanno anche beneficiato degli incentivi del conto energia. O ancora, gli incentivi per gli impianti fotovoltaici collocati su discariche chiuse, cave esaurite, aree bonificate. Poi, siamo riusciti a farvi capire l'importanza di estendere a tutto il territorio nazionale gli incentivi ai giovani agricoltori prima previsti solo per il Sud, che permetterà un ricambio generazionale. E poi la sburocratizzazione per l'autorizzazione delle zone a carattere sismico, che rischiavano di essere condannate definitivamente a non essere ricostruite. Dicevo prima che questo decreto era una buona opportunità, ma su certi aspetti siete riusciti addirittura nell'impresa di peggiorare la normativa, anziché semplificarla. Prendiamo la rigenerazione urbana: le nostre città spesso si trovano con dei vuoti urbani da rigenerare, una necessità che non deve essere vista come speculazione, ma anzi come un'opportunità. Per togliere questi vuoti urbani bisognava incentivare chi vuole investire, non mettere paletti. Chi non ha un'esperienza sul campo come amministratore locale o come professionista, ma fa solo l'ambientalista *snob* da salotto, non si rende conto di cosa voglia dire trovarsi di fronte a edifici abbandonati, ricettacolo di balordi e delinquenza, che voi alimentate riempiendo le nostre città di clandestini. Se si vuole fare in modo che ci sia un consumo di suolo quasi pari a zero, si deve dare la possibilità di demolire e ricostruire all'interno del tessuto urbano, senza insuperabili vincoli burocratici. ho un capannone in una zona ormai residenziale, aspetto anni di pratiche e permessi e poi mi si dice che devo tenere gli stessi prospetti e le stesse sagome. Prendiamo esempio dalla rigenerazione urbana delle città europee, non restiamo legati al "non tocco nulla"; mettiamo dei paletti ben chiari sugli immobili vincolati e non in generale. Serve coraggio. C'è poi l'intervento sblocca-stadi. Permettetemi di ricordare alla senatrice Biti e al caro Matteo Renzi, che forse sono annebbiati dalla smania di visibilità e lo hanno dimenticato, che è stato approvato anche un nostro emendamento, ma soprattutto senza i voti della Lega, il loro emendamento non sarebbe passato vista la contrarietà dei loro alleati di Governo del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*. Questa è stata solo uno delle spaccature e dei mal di pancia all'interno della maggioranza. Siete piegati agli ordini della CGIL, come ha tranquillamente riferito in audizione un loro rappresentante, quando ha affermato di avere un proprio Gruppo parlamentare. E la CGIL è tutt'altro che semplificazione. *(Applausi)*. Ancora più evidente è stato l'ennesimo voltafaccia dei 5 Stelle: dall'uno vale uno e dallo *streaming* sempre e ovunque, si è passati a saldare la scatola di tonno che volevano aprire dopo aver sostituito però il tonno con una buona aragosta. Vi rendete conto di aver approvato un emendamento che permette di eliminare il dibattito pubblico dall'*iter* autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architetture di rilevanza sociale che hanno impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio? Ma voi non eravate i portavoce dei cittadini? O dopo esservi rinchiusi nella famigerata scatoletta di tonno pensate "chi se ne frega" del parere dei cittadini su TAV, TAP, termovalorizzatori e grandi infrastrutture? Come dicevo all'inizio, era una grande opportunità che avete colto solo in parte, o anche meglio soprattutto grazie al nostro contributo che ha migliorato il decreto. Purtroppo vi siete intestarditi su diversi articoli e invece di semplificare avete aumentato la burocrazia. Non è complicando le norme che si evita il malaffare, anzi è il contrario. Ci voleva più coraggio, più fiducia negli italiani e negli amministratori locali. Invece avete preferito prestarvi ad essere usati da chi ha come ideologia proprio la complicazione, il boicottaggio della libera libera iniziativa e la tortura burocratica verso cittadini e imprese. Mettendo la fiducia, il giudizio sul decreto da tecnico diventa politico e questo non era quello che volevamo. Il voto della Lega-Partito Sardo d'Azione sulla fiducia sarà quindi convintamente contrario.

per comprendere l'importanza di questo provvedimento, il decreto semplificazioni, bisogna volgere lo sguardo verso l'obiettivo finale, verso il futuro. Questo futuro e questo obiettivo corrispondono ad uno dei punti più significativi che sono stati conseguiti da questo Governo grazie allo stimolo e al supporto continuo del MoVimento 5 Stelle. Tale obiettivo finale è rappresentato da un numero: 209 miliardi di euro. Si tratta di un grande piano di investimenti che noi potremo affrontare in questo Paese grazie al *recovery fund*, oramai ribattezzato Next generation EU, e non grazie alle operazioni di *marketing* o al piano *shock* evocati prima. Sul punto, però, credo sia importante fare una digressione: nel periodo più duro per il Paese, quello dei primi provvedimenti di chiusura delle attività produttive, la risposta dell'Unione europea è stata subito deficitaria. Nessuno di noi deve dimenticare che in quel momento era stato messo in campo un pacchetto che, prevedendo poche risorse date in prestito il piano SURE, la BEI o il MES, risultava del tutto inadeguato e non all'altezza dell'importante sfida davanti alla quale noi oggi ci troviamo. Ed è stato allora che che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sostenuto dall'impegno costante del MoVimento 5 Stelle, ha portato l'Italia a farsi capofila di otto Paesi per chiedere all'Unione europea una svolta, un cambio di passo, che mettesse in campo molte più risorse da reperire finalmente attraverso una massiccia e direi storica emissione di debito comune. Ed è esattamente quello che è successo: un'Europa finalmente diversa. Non ancora completamente quella che piace a noi, ma che sicuramente ha mostrato di poter recuperare quel valore della solidarietà di cui tanto abbiamo bisogno. Da qui arrivano i 209 miliardi messi a disposizione dell'Italia attraverso il *recovery fund*, di cui 80 miliardi in termini di sussidi. Mai, negli ultimi cinquant'anni, nel nostro Paese abbiamo avuto l'opportunità di realizzare un piano di investimenti nel digitale, nella transizione energetica, nell'ambiente, nel potenziamento e e completamento delle infrastrutture. Mai! Tutti questi punti, nessuno escluso, sono gli storici obiettivi che il MoVimento 5 Stelle è stato in grado di imporre all'Europa intera. *(Applausi)*. Ed eccoci arrivati al punto: non possiamo permetterci tentennamenti nella realizzazione di investimenti così ingenti. Abbiamo il dovere, nei confronti degli italiani, di mettere a terra rapidamente questi soldi e di dare una prospettiva di sviluppo alle nostre comunità Per tale ragione il decreto semplificazioni è fondamentale. Ci consentirà di sveltire e fluidificare tutta una serie di procedure senza abbandonare mai gli ineliminabili presidi a tutela della legalità e dell'ambiente. Questo decreto è stato davvero un grandissimo lavoro per tutti noi. Ricordiamolo: 2.900 gli emendamenti arrivati; oltre 1.000 quelli giudicati inammissibili; alla fine, saranno quasi 320 quelli approvati. Qui, il mio ringraziamento va ai due relatori, ai Presidenti delle Commissioni affari costituzionali e lavori pubblici, alla presidente Casellati e agli uffici di supporto. Il mio ringraziamento va anche ai colleghi delle opposizioni. Grazie al lavoro svolto in questi nove giorni, di cui molto in sedute notturne, abbiamo avuto la possibilità, insieme, di poter prevedere delle misure da realizzare per il bene del Paese. L'auspicio è che questo modo di collaborare possa proseguire anche in forma ordinaria, successivamente. I ringraziamenti, ovviamente, vanno anche ai Sottosegretari e al Governo, sempre presenti.

per proteggere il nostro tessuto economico produttivo ma, allo stesso tempo, per tracciare la strada di un pronto rilancio dell'economia. Parliamo di un decreto che porta avanti un'operazione di semplificazione amministrativa senza precedenti, inserendosi, peraltro, in perfetta linea di continuità con il decreto sblocca cantieri, condotto in porto durante il primo Governo Conte. Come dimostrato dal rapporto Cresme, il decreto sblocca cantieri stava dando dei grandi frutti, che potremo continuare a cogliere con il *recovery fund*. È grazie al decreto sblocca cantieri, infatti, che nel 2019 si è segnato un più 40 per cento delle emissioni di bandi pubblici per per quanto riguarda la concessione di lavori pubblici in questo Paese. E se andiamo a focalizzarci sui soli lavori pubblici, l'incremento è stato di oltre il 50 per cento. Ma noi sappiamo bene che non sono i bandi pubblici che ci consentono di spendere soldi nel Paese. Ecco perché stiamo intervenendo con il decreto semplificazioni, migliorandolo in sede di conversione. Come lo stiamo facendo? Con le procedure di aggiudicazione, che stiamo velocizzando con le procedure negoziate. Per gli affidamenti diretti siamo stati ad ascoltare la voce dei professionisti e di chi svolge servizi di ingegneria, architettura e di fornitura, abbassando la soglia che precedentemente era stata prevista dal Governo, portandola da 150.000 appunto a 75.000. Questo lo facciamo, però, senza mai derogare al principio della rotazione e della trasparenza, per noi cardini fondamentali. Fatemi inoltre dire, colleghi, che la semplificazione è un risultato cui dovremmo tendere con sempre maggiore intensità e convinzione. Come infatti sostengono tutte le Autorità indipendenti, è nelle lungaggini burocratiche che si annidano i più pericolosi rischi di inefficienze, opacità, incrostazioni affaristiche e infiltrazioni criminali. Su questo, quindi, rispediamo seccamente al mittente le accuse di aver abbassato la guardia. Insinuazioni tanto più risibili se consideriamo che, grazie al MoVimento 5 Stelle, questo Paese, con la legge spazza corrotti, si è dotato di presidi più all'avanguardia nel contrasto ai furbi e furbetti vari. Il decreto semplificazioni incide nella quotidianità, non soltanto nelle opere, come ricordavano alcuni colleghi delle altre forze politiche in precedenza. Nella quotidianità nel rapporto con i cittadini, sarà l'attuazione della Piattaforma digitale nazionale dati che ci consentirà di realizzare l'obiettivo che è il *once only*; quell'obiettivo per cui il cittadino una sola volta deve produrre un certificato o un documento alla pubblica amministrazione. E se un'altra pubblica amministrazione vuole lo stesso documento dall'impresa o dal cittadino, lo va a chiedere all'altra pubblica amministrazione e non nuovamente al cittadino. Potenzieremo i servizi attraverso la *app* IO, ricordata prima anche dalla senatrice Mantovani, con la quale potremo avere più facilmente autocertificazioni e formulare istanze. Sostituiremo la raccomandata cartacea con la comunicazione digitale ed i cittadini avranno finalmente l'accesso a tutti i servizi, grazie allo SPID e alla carta d'identità elettronica. Anche nella ricalibratura dell'abuso d'ufficio e della responsabilità erariale non c'è nessun passo indietro o colpo di spugna. Quanto all'abuso d'ufficio, prevediamo che, per configurare l'illecito da parte del pubblico ufficiale, non si dovrà più tenere conto dell'eventuale violazione di generiche norme di legge o di regolamento, ma della violazione di

L'attuale formulazione è troppo ampia e generica e, spesso, genera immobilismo per paura di infrangere le norme. Allo stesso tempo, come dicevo, rivediamo il tema della responsabilità erariale, in modo tale da contrastare il fenomeno della paralisi della firma da parte dei funzionari pubblici. Per questo prevediamo di mantenere una responsabilità erariale più grave in caso di comportamenti omissivi da parte dei funzionari stessi. In sostanza, la responsabilità erariale del funzionario che agisce - e cioè che firma - viene limitata alla sola ipotesi di dolo, mentre resta per dolo e colpa grave in presenza di omissioni. Abbiamo cercato di semplificare anche la procedura in tema di lavori edili privati. Abbiamo ridotto i tempi per l'autorizzazione sismica o, piuttosto, inizio attività (SCIA), anziché al permesso a costruire, nel caso anche di variazione di prospetti, per quegli interventi di demolizione e ricostruzione nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma del 2016. Non è affatto vero, infine, che l'intervento blocca la rigenerazione urbana nei centri storici, che invece viene ben codificata con l'estensione degli ambiti di tutela dai soli centri storici anche alle zone assimilabili alle zone omogenee A e a quelle di particolare pregio storico e architettonico. Presidente e colleghi, il Paese ha di fronte a sé una storica occasione. Le ferite lasciate aperte dal Covid e il tragico prezzo pagato in termini di vite umane resteranno per sempre nella nostra mente, ma dobbiamo far sì che convivano con il ricordo dell'enorme impegno profuso per cambiare un Paese che finalmente sarà tornato a correre.

del Gruppo Misto. Ognuno di noi, quando sente parlare di semplificazione, non può che ben sperare e ciò vale anche per ogni cittadino e ogni imprenditore e per chi è impegnato nelle file dell'amministrazione pubblica. Come IDEA e CAMBIAMO, dunque, eravamo ben disposti su questo fronte. D'altronde, l'idea che sia necessaria un'amministrazione pubblica che sappia semplificare le proprie procedure per dare in tempi ragionevoli risposte concrete ai bisogni del Paese è uno dei tratti che caratterizzano la nostra visione politica. Dopo che lo abbiamo urlato in ogni sede, pare che l'esigenza di semplificare e di innovare sia diventata evidente a tutti, persino a questo Governo. Purtroppo, come temevamo, le proposte nate dall'Esecutivo e dalla maggioranza sono solo una serie male articolata di interventi emergenziali, transitori e sperimentali che non guardano al sistema e ai processi nel loro complesso e che rischiano di creare un quadro regolatorio che complica anziché semplificare. A questo è necessario aggiungere che la maggior parte delle proposte avanzate dalle opposizioni e da Cambiamo, in particolare, non sono state ascoltate. Al di là di una serie di promesse, che poi bisognerà saper realizzare e naturalmente vedremo se ci riuscirete - purtroppo in questo provvedimento mancano una visione complessiva e la capacità di darle una declinazione organica e puntuale. Rischiamo dunque di approvare un disegno di legge complicazioni e non semplificazioni e per questo il nostro voto sarà assolutamente contrario.

sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

(c'è un assembramento improbabile).

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.900, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, e acquisita la relazione tecnica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: siano soppresse le previsioni di cui agli emendamenti

Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguente modifiche: all'emendamento 7.7 (testo 2), al comma 7-*ter*, sostituire le parole: "a decorrere dall'anno 2021", con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022" all'emendamento 8.69 (testo 2), alla lettera *c)*-*ter*, sostituire le parole: "gli enti territoriali possono" con le seguenti: "gli altri enti pubblici territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"; all'emendamento 37.1 (testo 2), sia aggiunto, infine, il seguente comma: "2-*bis.* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare

l'emendamento 39.0.39 sia sostituito dal seguente: "All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio *(venture capital*) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.A., mediante apposita convenzione. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente comma."; all'emendamento 40.0.14 sia aggiunto, infine, il seguente comma: "2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."; all'emendamento 43.0.98, il comma 3 sia sostituito dal seguente: "All'attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."; all'emendamento 48.20 (testo 2), al comma 7-*bis*, siano aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente provvede, ove necessario, ai conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica."; all'emendamento 49.0.22, al comma 2 sia soppresso l'ultimo periodo e sia aggiunto, infine, il seguente comma: "3. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."; all'emendamento 62.0.2, il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. ("SFBM") subconcessionaria del soggetto di cui al decreto riportato nel presente comma, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145."; al medesimo emendamento 62.0.2, al comma 4, dopo le parole: "con decreto del Ministero dello sviluppo economico", siano inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze"; all'emendamento 62.0.5 (testo 3), al comma 1, sostituire le parole: "produzione annuale da esse ottenuta", con le seguenti: "produzione da esse ottenuta nell'anno precedente.".

con appello. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto,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

e

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 76.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

Ho sempre considerato il mese di settembre un po' come il primo gennaio, dove si cerca di tirare le somme dei mesi passati e si fanno i buoni propositi per il nuovo inizio. Guardandoci alle spalle, abbiamo trascorso dei mesi molto pesanti sofferenze, crisi economiche, perdite di tutti i cittadini che hanno pagato il prezzo di questa pandemia, chi con il lavoro, chi addirittura con la vita. Con l'arrivo dei mesi estivi, tutti volenterosi e pronti alla rinascita, abbiamo voluto investire sulla fiducia nei cittadini, premiarci dopo i mesi di *lockdown* e tentato di far ripartire l'economia con il turismo. Penso naturalmente alla mia isola che a giugno veniva definita Covid *free*, che ha raggiunto oltre 7 milioni di presenze, nonostante il periodo sicuramente non favorevole, e si è rivelata, ancora una volta, meta preferita dagli italiani e non solo. All'inizio dell'estate noi sardi eravamo però titubanti, conoscevamo i rischi che avremmo corso nell'essere una destinazione così gettonata e, di conseguenza, per tutelarci, abbiamo proposto il certificato di negatività, venendo sbeffeggiati dal Governo e paragonati alla Corea del Sud. Mesi dopo, quando l'estate volge alla sua fine, dopo che milioni di italiani si sono riversati sulle spiagge della mia isola, vediamo le naturali e ovvie ripercussioni sanitarie date dalle misure non adatte imposte dal Governo. Vediamo anche una campagna mediatica strumentalizzata dalla sinistra, che fa passare la Sardegna come isola di untori, quando l'unica cosa che siamo stati è vittime vittime di un Governo non curante, che ha preferito pensare alle proprie poltrone piuttosto che assecondare la richiesta del presidente Solinas ed evitare tanti contagi inutili. Non c'è stata alcuna negligenza da parte della regione Sardegna ed è inutile il *dossier* che la Giunta Zingaretti ha presentato al ministro Speranza per denunciare la mancata collaborazione dell'isola dopo l'impennata dei contagi. Nel mese di luglio la Sardegna aveva lo 0,3 di sieroprevalenza un dato certificato dal Ministero della salute. Così come ha dichiarato il presidente Solinas, la responsabilità di controllare la salute di chi passa le frontiere e si muove negli scali è del che attraverso gli uffici sanitari di frontiera... *(Il microfono si disattiva automaticamente)* ...deve assumersi queste responsabilità. Quindi è inutile dire che i casi positivi, che si registrano nel Lazio, provengono dalla Sardegna per negligenza della Regione; piuttosto si è saputo dai giornali, da molte testimonianze e dai *social network* che molti giovani, pur di passare indenni ai controlli, assumevano paracetamolo. Dunque, non credo proprio che questa responsabilità possa essere attribuita alla nostra isola. Come dicevo all'inizio del discorso, colleghi, settembre è un mese in cui bisogna guardare avanti e pensare ai buoni propositi. Mi auguro dunque fortemente che le persone che si sono permesse di condannare la mia isola, si facciano un esame di coscienza, come per esempio il governatore Zingaretti, che è stato il primo a pagare le conseguenze della sua negligenza nei confronti della pandemia, passando dagli aperitivi in Corso Como al suo isolamento nel mese di marzo. Smetta di puntare il dito contro il governo sardo, ma cerchi di trovare un modo costruttivo per affrontare la situazione. La pandemia si può sconfiggere solo…

Intanto però il governatore della Sardegna, Solinas, ha dato mandato ai legali della Regione di valutare il reale danno della campagna mediatica, poiché continuano ad arrivare disdette e, soprattutto, si è presentata una situazione che è di assoluta falsità. **Atti e documenti,